Colleghi, vi inviterei a un minimo di silenzio e di compostezza perché non si riesce neppure a sentire quello che legge il senatore Segretario.

nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché del parere della Giunta per il Regolamento, espresso nella seduta del 7 giugno 2006, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella Regione Lombardia, a seguito delle dimissioni del senatore Roberto Formigoni, ha riscontrato nella seduta odierna che il candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo della lista alla quale apparteneva il predetto senatore è Riccardo Conti. Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e proclamo senatore Riccardo Conti. Avverto che da oggi decorre nei confronti del nuovo proclamato il termine di 20 giorni per la presentazione di eventuali reclami.

recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee;

precisato - credo che sia opportuno ribadirlo - che non incombono pericoli di sanzioni o di risarcimenti danni miliardari (com'è stato anche chiarito in un intervento),

Abbiamo ascoltato dal senatore Butti di alcune storture e abusi sostanziali, sia pure compatibili con la legge, che ci sono attualmente: anche su questi bisognerà intervenire. Prendo però atto con soddisfazione che, anche da parte di senatori senatori dell'opposizione, è emerso un giudizio almeno parzialmente positivo sull'articolo 8*-novies*, giudicato da alcuni non sufficiente, ma comunque un passo avanti. Credo sia quanto si poteva fare in questa circostanza, quella di un decreto-legge Per quanto riguarda le colleghe Bonino e Adamo, intervenute sull'articolo 8*-duodecies*, ricordo

Voglio cogliere, in particolare, l'esortazione del senatore Santini alla ratifica del Trattato di Lisbona, che evidentemente è il quadro che tiene tutta questa normativa. Ringrazio anche il senatore Mazzatorta per aver richiamato gli effetti pratici

adeguare le nostre leggi alle normative europee, a ricordare che queste ultime non sempre hanno solo riflessi positivi, ma possono mettere in grave difficoltà taluni soggetti. Anche in questa

erano molto più pacati di quanto fossero in esordio della discussione del noto emendamento che abbiamo introdotto nel decreto cosiddetto salva-infrazioni. In molti interventi

di alcuni numeri inerenti al problema delle frequenze. Molti hanno detto e sostenuto, sia questa mattina che alla Camera la scorsa settimana, ma anche nelle polemiche che accompagnano nel Paese tutte le materie che riguardano la televisione, che due operatori

che emerge un dato profondamente diverso da quello che più di una volta polemicamente si sostiene sia. Siccome nell'emendamento si fa anche cenno alla procedura utilizzata in Sardegna

da un regime analogico ad un regime digitale, in Sardegna ci saranno 2 multiplex che il Ministro potrà attribuire. Quindi, si tratta della bellezza di 10 canali. Siccome ho sentito alcuni accenni critici questa mattina, ma anche nei giorni scorsi, sulla procedura che è stata utilizzata in Sardegna, voglio solo sommessamente ricordare ai colleghi del Partito Democratico che nel loro programma c'è scritto che «i criteri di proporzionalità, non discriminazione, trasparenza e apertura a nuovi entranti che sono stati adottati per la transizione in Sardegna» - sto citando il programma del Partito Democratico - «saranno alla base della transizione nazionale».

a mio avviso un po' inventate, sul famoso periodo che è stato poi eliminato. Perché lo avevamo inserito? Perché nel Codice delle comunicazioni, all'articolo 28, si dice letteralmente: «Al fine di agevolare la conversione del sistema dalla tecnica analogica alla tecnica digitale (...) prosegue con l'esercizio degli impianti di diffusione e di collegamento legittimamente in funzione alla data di entrata in vigore»,

potuto essere attivate, in questo caso ci ha detto che non le basta sapere che funzionino, ma che vuole avere una data di chiusura, di cessazione, e questo è quello che era stato fatto; fatto; nel periodo, che poi è stato eliminato perché su di esso si è innestata una polemica politica assolutamente pretestuosa, era stata messa, con definizione identica a quella che ho appena citato al comma 1 dell'articolo 28, una data di chiusura e di cessazione degli impianti. impianti. Francamente quindi non abbiamo capito, ma abbiamo accettato che la polemica politica in questo caso non ci consentisse di portare avanti quel ragionamento ed abbiamo consentito di togliere questo periodo.

di licenza ad un regime di autorizzazione, il che vuol dire, in parole povere, che chiunque faccia una DIA, una dichiarazione di inizio attività, ha l'autorizzazione a trasmettere, quindi non è più un titolo abilitativo con valore di licenza, ma è un titolo di autorizzazione generale. Questo consente di risolvere il secondo problema che ci veniva contestato dall'Europa, quello dell'accesso a quello che viene chiamato in gergo tecnico il *trading*, cioè il mercato delle frequenze: chiunque può accedere al mercato delle frequenze e non ha questa barriera all'accesso che l'Europa non ci consentiva di avere. Ma il passaggio più importante (su questo il senatore Vita, a mio avviso,

Quindi, non assume il Ministero o il Ministro o il Governo una gestione diretta delle frequenze, ma definisce solamente un calendario in base ad un piano di attuazione che rimane per intero alla Agcom; si consente in

ma probabilmente di stimolare un percorso nelle Regioni più importanti e di fare in modo che nell'arco del 2009, 2010, forse 2011, molte Regioni italiane possano passare da un regime analogico ad un regime digitale. Questo è il senso complessivo dell'emendamento che abbiamo inserito nel decreto-legge, ovviamente parlo solo per la materia di mia competenza, ma mi sembrava che su questo punto almeno vi potesse essere un accordo complessivo. L'Europa ci ha fatto alcune domande, abbiamo dato velocemente e concretamente alcune risposte, abbiamo usato un vettore legislativo veloce come può essere quello del decreto-legge e su questa base oggi siamo in grado di dire all'Europa che su questi tre punti (non quattro come avremmo voluto) abbiamo dato una risposta. Tutto questo per evitare che l'Europa, la Commissione europea, in particolare il commissario Kroes, che è già arrivata al secondo grado della procedura d'infrazione, cioè al parere motivato, eviti di passare al terzo grado, che è quello del deferimento alla Corte di giustizia.

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza in relazione al testo, testo, parere di nulla osta, nel presupposto che, come affermato dal Governo, le convenzioni di cui all'articolo 8-*duodecies* non producono effetti finanziari diretti per la finanza pubblica né sul bilancio dell'ANAS. Rileva, inoltre, la necessità di un rispetto rigoroso delle procedure di verifica parlamentare in relazione alle successive modificazioni o integrazioni delle Convenzioni. Ritiene inoltre necessaria l'acquisizione degli atti relativi alle concessioni approvate di cui al comma 2. Esprime, infine, parere di semplice contrarietà sull'articolo 5. Per quanto concerne gli emendamenti, esprime parere non ostativo ad eccezione delle proposte 8-*duodecies*.2, 8-*duodecies*.3 e 4-*bis*.0.1, sulle quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

la norma recata dall'articolo 8-*duodecies,* relativo alle concessioni autostradali, presenti gravi problemi di scorretta copertura e quindi di mancato rispetto dell'articolo 81

è perfettamente parte del perimetro delle pubbliche amministrazioni. Negli anni scorsi, si è sviluppato un tentativo (in Italia per l'ANAS, in Germania per altre società) le società volte alla realizzazione di infrastrutture dal novero delle pubbliche amministrazioni. Questo tentativo si è concluso con una decisione della Commissione europea che ha riaffermato, con grande nettezza, che intanto una società di questo tipo può uscire dal novero delle pubbliche amministrazioni in quanto almeno il 50 per cento dei suoi proventi derivi da iniziative sviluppate sul mercato. Non essendo questo patentemente il caso dell'ANAS, quest'ultima è quindi perfettamente parte del perimetro delle pubbliche amministrazioni.

il recupero della parte degli introiti tariffari relativi a impegni di investimento programmati nei piani finanziari e non realizzati nel periodo precedente. Tradotto dal politichese delle leggi, in buona sostanza, se un concessionario autostradale si era impegnato a realizzare investimenti che non ha realizzato totalmente, quando si rinnova la concessione, il concedente, cioè l'ANAS, interviene per fare in modo che le tariffe vengano modificate, e vengano quindi imposti obblighi sul concessionario, in modo tale che l'obbligo alla realizzazione degli investimenti venga perfettamente rispettato. In caso contrario, è del tutto evidente cosa accade: vengono imposte sugli automobilisti e sui camionisti delle tariffe giustificate dalle politiche di investimento che poi non si realizzano, consentendo un sovrapprofitto del tutto illegittimo alle società concessionarie. Signor Presidente, siccome si va ad un rinnovo al buio per il Parlamento di queste concessioni, tali norme, che ricadono perfettamente tra quelle che incidono sul bilancio dell'ANAS, che fine fanno? La Corte dei conti ha lanciato un allarme molto serio su questo punto quando ha detto che l'ANAS è parte delle pubbliche amministrazioni; quindi, quando si determinano oneri a carico dell'ANAS, si determinano oneri a carico della pubblica amministrazione. Di conseguenza, questa norma, che cancella la procedura in vigore sul versante delle concessioni per affermarne una nuova con il rinnovo *ope legis*, è stata criticata per l'aspetto meno rilevante, cioè per il fatto che sarebbe un intervento *ope legis*. Il problema non è questo; il problema è che si modifica la legislazione vigente a danno dell'ANAS e a favore dei concessionari senza intervenire con la necessaria copertura.

Nel frattempo, forse per accrescere l'attesa del provvedimento Robin Hood, ha consentito che si facesse un provvedimento come questo, sceriffo di Nottingham, nel quale lo sceriffo di Nottingham sono le concessionarie, i poveri contadini tartassati

Senatore Morando, la Presidenza prende atto delle sue osservazioni, ma le ricorda che non può fare a meno del prendere atto anche del parere espresso dalla Commissione bilancio, per cui

che adegua in via interpretativa alcune disposizioni regolanti la funzione di risanamento del dissesto finanziario dell'ente ospedaliero Ordine Mauriziano, affidate alla fondazione Ordine Mauriziano, adegua ai princìpi fissati dalle norme sovranazionali. Costituisce pertanto attuazione di obblighi di rispetto della disciplina comunitaria in materia; da qui la richiesta di introduzione di tale articolo all'interno del provvedimento in esame.

dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, aveva istituito la fondazione Ordine Mauriziano trasferendo alla fondazione medesima il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'ente Ordine Mauriziano allo scopo di gestire il patrimonio e i beni trasferiti e di operare per il risanamento del dissesto finanziario dell'ente stesso, anche mediante la dismissione dei beni del patrimonio disponibile trasferito, ad eccezione dei presidi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro (IRCC) di Candiolo (Torino), poi inseriti nell'ordinamento sanitario regionale. Il comma 3 del medesimo articolo 2 ha disposto la successione della fondazione nei rapporti attivi e passivi e nelle situazioni debitorie e creditorie a qualsiasi titolo maturate dall'ente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, esclusi i rapporti di lavoro relativi alle attività sanitarie. Il comma 1350 dell'articolo 1 della legge finanziaria del 2007 ha chiarito come restino esclusi dal trasferimento alla fondazione Ordine Mauriziano i beni immobili e mobili (l'ospedale Umberto I) o mobili (Istituto di ricerca sul cancro di Candiolo), funzionalmente connessi allo svolgimento delle attività istituzionali dei presidi richiamati. In considerazione della situazione di dissesto finanziario della stessa fondazione Ordine Mauriziano, l'articolo 30 del decreto-legge n. 159 del 2007, convertito poi con la legge legge n. 222 del 2007, ha provveduto al commissariamento della fondazione Ordine Mauriziano. La scissione del patrimonio dell'ente, operata dagli articoli 1 e 2 del citato decreto-legge n. 277 del 2004 confermata dal comma 1350 dell'articolo 1 della legge finanziaria del 2007 se, da una parte, disciplina il diverso regime della titolarità dei beni tra soggetti giuridici subentranti all'ente Ordine Mauriziano non può, dall'altra parte, comportare la sottrazione al patrimonio della fondazione del corrispettivo, da determinare ai valori di mercato, di una cospicua parte dei beni già di proprietà dell'Ordine Mauriziano, che la stessa legge ha destinato al soddisfacimento dei creditori dell'ente Ordine Mauriziano. Una diversa interpretazione delle norme che di ciò si occupano si porrebbe, infatti, in contrasto con l'articolo 42 della Costituzione, determinando un'illegittima lesione dell'autonomia patrimoniale della fondazione, posta dalla legge istitutiva della fondazione medesima, a garanzia dei creditori dell'ente, secondo quanto previsto dall'articolo 2744 del codice civile. A tale riguardo, occorre tenere presente che da un creditore dell'ente Ordine Mauriziano è già stata sollevata questione di illegittimità costituzionale

348 e 349 del 2007) in materia di determinazione delle indennità di espropriazione, ha affermato che la perdita del diritto di proprietà, cui nella fattispecie è riconducibile la perdita della garanzia dei creditori su una parte significativa del patrimonio dell'ente debitore insolvente, non può avvenire senza un ristoro economico che non corrisponda al valore reale del bene. Quindi, l'articolo che si propone vuole fornire un'interpretazione maggiormente coerente con il dettato costituzionale delle norme sopra citate, chiarendo che i corrispettivi dei beni immobili e mobili, separati dal patrimonio trasferito alla fondazione e rimasti all'ente ospedaliero e calcolati ai valori di mercato, confluiscono nella massa attiva destinata alla soddisfazione dei creditori concorsuali dell'ente medesimo.

intende illustrato.

qual è lo stato dell'arte nel recupero delle frequenze ridondanti da attribuire in base alla sentenza della Corte di giustizia europea, e da ultimo il Consiglio di Stato,

propone di sopprimere il comma 2 dell'articolo 8-*duodecies*, introdotto dalla Camera dei deputati su proposta del Governo, il quale dispone l'approvazione *ex lege*, in luogo di quella amministrativa, di tutti gli schemi di convenzione con la società ANAS spa già sottoscritti dalle società concessionarie autostradali alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame. Si tratta di un caso tipico di legge‑provvedimento con cui vengono sottratte alle procedure vigenti, sia per quanto concerne l'*iter* approvativo in senso generale, sia per quanto concerne la fase di valutazione contabile in senso stretto, determinati schemi di convenzione tra società concessionarie e ANAS spa. Occorre dunque valutare con particolare attenzione la portata e gli effetti di questo trasferimento dalla sede amministrativa a quella legislativa del momento approvativo finale, avendo bene presente che avverso le disposizioni legislative non sono esperibili i rimedi tipici dei provvedimenti amministrativi e che, al contempo, altri schemi di convenzione sono stati depositati. Ritengo pertanto necessario richiamare all'Assemblea le disposizioni vigenti che vengono derogate dal decreto-legge in esame. ha novellato il testo dei commi 82-89 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, dettando più rigorose disposizioni sul procedimento di esecuzione degli accordi tra ANAS e subconcessionarie.

sono conseguiti ai sensi dell'articolo 2, comma 84, del decreto-legge n. 262 del 2006, laddove si stabilisce che gli schemi di convenzione unica, sentiti il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), le associazioni rappresentative delle società concessionarie e quelle di consumatori e utenti, siano sottoposti dapprima all'esame del CIPE e successivamente alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Si era inteso in tal modo porre rimedio in via legislativa alle lacune delle convenzioni in essere in fatto di adeguate clausole a salvaguardia degli interessi della collettività. Intervenendo su tale quadro, l'articolo 8-*duodecies* dispone che tale procedura complessa venga sostituita con la validazione immediata per via legislativa degli schemi di convenzione che sono attualmente in corso di approvazione. Va innanzitutto rilevato come l'articolo aggiuntivo, approvato nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, risulti sprovvisto di relazione tecnica per quanto concerne gli effetti finanziari, ma preme soprattutto segnalare i suoi effetti sulla trasparenza delle condizioni di affidamento delle concessioni autostradali, problematica rilevata anche dal Servizio studi del Senato. La rinuncia agli adempimenti procedurali e ai controlli che la legge impone di effettuare prima della definitiva approvazione degli schemi comporta anche la preventiva trasmissione degli schemi di convenzione alle Camere, per il parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, ma anche per le conseguenze di carattere finanziario. Vi è quindi la possibilità di effetti onerosi per l'erario aggiuntivi a quelli ipotizzabili, attualmente non valutabili, dal momento che le Camere non verranno più investite di un dovere-diritto di valutazione sugli schemi, con particolare riferimento per il recupero della parte degli introiti tariffari relativi a impegni di investimento programmati nei piani finanziari e non realizzati nel periodo precedente, dinamica dei costi, tasso di efficienza e qualità conseguibile dai concessionari e altro ancora. Si tratta di aspetti che chiamano in causa il soggetto titolare della potestà concessoria,vale a dire l'ANAS, la quale, ancorché soggetto formalmente in regime di diritto comune ai fini giuridici, è da considerare amministrazione pubblica ai fini della contabilità nazionale. L'introduzione nel decreto in esame del comma 2, con la conseguente deroga alle consuete procedure di approvazione degli schemi che esso comporta, costituisce a nostro avviso un fattore di contrarietà ai princìpi contabili e di buon andamento della pubblica amministrazione, prefigurando inoltre un'ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni analoghe che pone seri dubbi sulla non manifesta irragionevolezza della norma stessa, privando inoltre le Camere della funzione di controllo attribuita dalla legge. anche tenendo conto del fatto che il primo comma dell'articolo aggiuntivo contiene disposizioni condivisibili, si raccomanda l'approvazione dell'emendamento soppressivo e, in ogni caso, l'accoglimento dell'ordine del giorno relativo alle informazioni che devono comunque essere rimesse al Parlamento per consentire la trasparenza e la conoscibilità delle procedure adottate e degli effetti che esse sono suscettibili di produrre.

a giusta ragione, obbligatorio richiamare i nostri doveri, tra cui quello di essere consapevoli al momento del voto e di conoscere appieno quelle che sono le proposte che vengono sottoposte all'Assemblea. *(IdV)*. Signor Presidente, onorevole colleghi, membri del Governo, lei ha ragione tanto più che quest'Aula ha applaudito fragorosamente gli studenti americani ai quali si sta oraimpedendo di ascoltare quanto viene detto.

L'emendamento poi sostiene che le emittenti che non sono state dotate delle frequenze necessarie per trasmettere devono essere dotate di questa potestà.

della normativa comunitaria o di decisioni di giudicato comunitario, ossia di sentenze della Corte di giustizia europea, perché lo strumento del decreto-legge non consente al Parlamento di valutare fino in fondo la portata, il contenuto e l'entità delle decisioni comunitarie.

al dettato costituzionale, che solo il Parlamento può fare. Riteniamo quindi che lo strumento del decreto‑legge sia eccessivo e non sia neanche giustificato dalla necessità di anticipare i tempi dell'esecuzione di una sentenza degli organi di giustizia europea.

che non sono interessati ad ascoltare le dichiarazioni di voto ad astenersi dal brusìo o a lasciare l'Aula, perché il senatore D'Alia ha il diritto di esprimere la sua dichiarazione di voto

arretrando rispetto a valutazioni sul contenuto che certamente anche il decreto-legge avrebbe meritato. Questa è un'altra ragione per la quale siamo contrari.

che riteniamo grave la circostanza - in linea di principio, ma anche sotto il profilo del merito del provvedimento - che si possa per legge approvare bozze di schemi di convenzioni autostradali

almeno un impegno politico da parte del Governo a sottoporre questi atti e provvedimenti ad un minimo di controllo e di informativa del Parlamento. Tutto ciò incide negativamente sulla qualità e sulla quantità, ad esempio, delle manutenzioni e degli investimenti che, in questo settore, sono fondamentali e strategici. Viene meno, quindi, quella parte che riteniamo essenziale in un rapporto concessorio, che è il controllo pubblico. Quest'ultimo viene effettuato non perché la mano pubblica debba sostituirsi al privato concessionario, ma per garantire gli interessi pubblici sottesi ad una concessione, cioè l'interesse generale ad un migliore e più efficiente funzionamento del settore.

quindi, un sistema che, proprio per la natura dello strumento legislativo utilizzato - cioè la decretazione d'urgenza - blinda un provvedimento, senza dare al Parlamento alcuna possibilità di effettuare verifiche e controlli. È un precedente - non il solo, per la verità, perché ve ne sono tanti molto grave. Se riteniamo, infatti, che il processo di devoluzione dell'ordinamento comunitario - e, quindi, il recepimento nel nostro Paese delle direttive, dei regolamenti comunitari e delle decisioni giudiziarie europee sia un meccanismo che può essere affidato ad un decreto-legge e non agli strumenti rodati (come le leggi delega e quant'altro), introduciamo uno strumento surrettizio che non consentirà al Parlamento di recepire il 70 per cento della normativa comunitaria, soprattutto di quella che ha rilievo ed importanza per tutti i settori

nuova modifica della disciplina sull'emittenza e sull'uso delle frequenze, è la testimonianza, forse in tono minore, di una politica che si è affermata instancabilmente negli ultimi due decenni e che dal 1994 si configura, né più né meno, come una sorta di uso privatistico dello Stato. Le imprese del titolare di un impero delle comunicazioni private, che nel frattempo si è ritrovato ad essere un protagonista della scena politica, vengono sistematicamente protette,

La cosa è tanto più evidente quando addirittura si vede che a piccole emittenti televisive, che non potrebbero portare nocumento di sorta ad un grande impero,

costantemente ad una politica che tende a proteggere le imprese di cui è titolare, di volta in volta, il Presidente del Consiglio o il capo dell'opposizione senza senza tenere nel giusto conto gli inviti, che vengono da più sedi istituzionali, al rispetto del pluralismo dell'informazione e della possibilità di una competizione in condizioni di parità per tutti i soggetti interessati. Questo è il motivo fondamentale per cui l'Italia dei Valori voterà contro questo provvedimento. Per gli altri argomenti si associa alle argomentazioni e alle motivazioni già addotte dai colleghi che sono intervenuti in precedenza.

Presidente, colleghe e colleghi, il provvedimento che stiamo per approvare e sul quale preannuncio il voto favorevole della Lega Nord interviene su temi molto diversi tra loro e ha carattere di urgenza, visto che deve adeguare le leggi dello Stato italiano ad obblighi comunitari la cui scadenza era anteriore alla legge comunitaria relativa all'anno in corso. Desidero tuttavia svolgere alcune considerazioni puntuali rispetto a taluni articoli del provvedimento ed altre considerazioni di carattere più generale. Non parlerò di frequenze televisive, perché penso che se ne sia già parlato anche troppo. Rispetto agli articoli 1 e 2, spero che ci rendiamo tutti conto che il recepimento della normativa è destinato a produrre, come è già stato detto dal collega Mazzatorta, gravi problemi per quelle aziende che in passato hanno ottenuto finanziamenti considerati aiuti di Stato e che ora, vista l'entità di tali trasferimenti e la richiesta di rientro immediato da parte di enti creditori (ad esempio l'INPS), rischiano il fallimento. La norma riportata all'articolo 6 6 è indispensabile per superare le procedure di infrazione, anche se potrebbe risultare penalizzante per i gestori di discariche che dovranno anticipare al primo ottobre 2008 la data di ultimazione dei lavori di adeguamento delle stesse, anche se i propri piani di adeguamento potrebbero prevedere tempi più lunghi. Rispetto all'articolo 8-*quater*, in linea con tali disposizioni la Lega Nord ha presentato un proprio ordine del giorno,

quella che volevano era un'Europa dei cittadini, non quella delle banche, delle *lobbies* e delle multinazionali. Un'Europa garante della pace, veramente democratica, dove i cittadini possano davvero dire la loro. Ricordo che l'unico organismo europeo votato democraticamente con suffragio universale (e questo - lo ricordo - avviene solo da meno di tre decenni perché prima anche i deputati europei erano semplicemente nominati) è il Parlamento europeo, che nei fatti (rispetto alla Commissione e al Consiglio) conta però pochissimo. I nostri cittadini conoscono così poco dell'Europa che la maggiore parte di essi immagina, al contrario, che (come nel nostro Paese) sia il Parlamento a legiferare. La disaffezione verso le istituzioni europee ha toccato il culmine con la bocciatura del Trattato sull'Unione europea da parte di Francia e Olanda, ma non so sinceramente cosa sarebbe successo se i cittadini degli altri Paesi avessero potuto esprimersi. Il problema di quest'Europa è che gli europei ne percepiscono solo il peggio. l'autoreferenzialità, le regole spesso intrusive che appesantiscono il già gravoso fardello burocratico che devono sopportare. Quest'Europa è cresciuta troppo velocemente. Forse sarebbe stato più saggio dilatare maggiormente nel tempo l'ingresso di nuovi Paesi nella Comunità, Paesi con problemi enormi che sicuramente si aspettavano molto di più di quello che potranno avere, almeno nell'immediato. nell'immediato. Sono convinta che l'Europa può e deve essere il motore per lo sviluppo dell'economia, della conoscenza, della sicurezza, ma se vogliamo che sia così allora dobbiamo convincere di questo i cittadini e non avere paura del loro giudizio. Se regole ci devono essere, devono essere regole condivise, chiare, non penalizzanti, utili agli europei. Il lavoro da fare è tanto, è necessario partecipare maggiormente e con maggiore determinazione alla costruzione di queste regole, magari impugnare qualche provvedimento di sanzione, come fanno altri Paesi della Comunità, quando la sanzione appaia ingiustificata o troppo penalizzante. Spero sinceramente che questo farà il nuovo Governo. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i senatori del Gruppo del Partito Democratico voteranno contro il provvedimento all'attenzione oggi dell'Aula del Senato. Il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, è stato infatti in punti essenziali stravolto, peggiorato da emendamenti della nuova maggioranza. Intendo riferirmi in particolar modo all'articolo 8-*novies* in materia radiotelevisiva e all'articolo 8-*duodecies* in materia di convenzioni delle concessioni autostradali. A noi dispiace prendere questa netta posizione di avversione, ma vi siamo costretti dalle decisioni assunte dalla maggioranza, che non solo non rispondono positivamente ed adeguatamente alla richiesta dell'Europa, ma riprendono, soprattutto in materia radiotelevisiva, la vecchia strada che antepone al diritto e agli interessi generali quelli di una parte. Il nuovo clima politico di dialogo e di confronto tra avversari non più nemici, nuovo clima politico a cui il Partito Democratico ha contribuito grandemente fin dalla sua nascita, avrebbe dovuto consigliare la maggioranza ad un atteggiamento più prudente in materia radiotelevisiva e, consentitemi, anche un po' più di stile in materie che per i nostri cittadini erano e restano materie eticamente e politicamente sensibili, perché coinvolgono princìpi di libertà economica, come mercato e concorrenza, e valori costituzionali quali il pluralismo e la libertà di informazione. Invece, il Governo Berlusconi, in modo un po' pavloviano, reagisce sempre allo stesso modo: prima gli interessi dell'azienda, poi gli interessi del Paese e le regole europee. Davvero speravamo in un altro esordio. Solo la tenace battaglia delle opposizioni alla Camera ha obbligato il Governo a cancellare dal provvedimento gli aspetti più inaccettabili, quelli che la stampa di ogni tendenza ha giustamente chiamato «salva Retequattro». Questa battaglia vinta ci consente oggi di ragionare più pacatamente e di approfondire meglio le ragioni del nostro dissenso, che rimane tale. Certo dispiace che non vi sia una adeguata sensibilità, sia dell'onorevole Romani, che ha parlato ed ora è assente, ma soprattutto del rappresentante del Ministero delle infrastrutture, che neppure ha sentito il bisogno di rispondere nell'Aula del Senato alle osservazioni poste dal dibattito. Quanto a stile, direi che oggi siamo veramente in ribasso. Ricordo brevemente le contestazioni della Commissione europea: l'esigere che le imprese ottengano una licenza individuale anziché una autorizzazione generale per la gestione di una rete di impianti; la limitazione della compravendita di frequenze alla trasmissione digitale e la possibilità per gli operatori di mantenere il controllo delle loro frequenze analogiche fino a dopo la data dello *switch off*, cioè della transizione definitiva al digitale; la mancata previsione di procedure trasparenti, eque e non discriminatorie per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze; il circoscrivere ai soli operatori analogici esistenti della possibilità di accedere alla sperimentazione di trasmissioni terrestri con tecnica digitale, alle licenze di operatore di rete digitale e alla compravendita delle frequenze; il conseguente impedimento per i nuovi operatori di installare e gestire una rete digitale e di acquisire o utilizzare frequenze per trasmissioni digitali; il consentire agli operatori analogici di convertire le proprie licenze analogiche (e quindi le proprie reti) in licenze digitali fino alla data dello *switch off* e senza restrizioni; la mancata limitazione del numero di frequenze acquisibili a quanto esattamente necessario per sostituire i loro attuali programmi analogici con programmi digitali, senza obbligo di restituire le frequenze liberate. Mi scuso per il tecnicismo, ma purtroppo questa è una materia molto tecnica ed è corretto che rimangano puntualmente agli atti del Senato quali sono i rilievi della Commissione europea, che sono stati poi accolti dalla Corte di giustizia europea. Queste sono le censure europee alle leggi italiane. A ciò l'articolo 8-*novies*, anche nella versione meno negativa approvata alla Camera dei deputati, non risponde o risponde in modo parziale. Non voglio tediare gli onorevoli colleghi con questioni che a molti possono apparire un po' esoteriche, ma mi corre l'obbligo di ricordare che la Corte di giustizia europea il 31 gennaio di quest'anno ha accolto gran parte delle tesi del giudice del rinvio e ha così ribadito che le norme italiane di assegnazione delle frequenze radiotelevisive non rispondono a criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati, richiesti dalle direttive europee. La sentenza ricorda che nemmeno l'intervento della Corte costituzionale ha consentito di risolvere la *vexata quaestio* dell'attribuzione delle frequenze. Infine, anche il Consiglio di Stato, con sentenza del 31 maggio 2008, che qui è stata ricordata in modo parziale se non distorto, relativa al caso Europa 7, ha chiesto al Governo di eseguire la sentenza europea sulle frequenze televisive, cioè di procedere all'assegnazione delle frequenze. È quello che chiediamo anche noi del Partito Democratico. In proposito, abbiamo presentato in primo luogo un emendamento che impegnava il Governo ad assegnare ai soggetti interessati le frequenze ridondanti e quelle che si liberano nel percorso di passaggio alla tecnica digitale, con criteri trasparenti e non discriminatori. Non è comprensibile che in tutto il mondo vi sia un dividendo digitale nel passaggio alla nuova tecnologia e solo in Italia questo non sia possibile. In secondo luogo, chiediamo al Governo un impegno per varare al più presto un disegno di legge finalmente in grado di armonizzare la legislazione italiana a quella europea e quindi rispondere nel merito alla sentenza della Corte di giustizia. Un disegno di legge capace di definire in modo organico il passaggio al digitale, valorizzando il mercato e la concorrenza che, non dimentichiamo, sono la *condicio sine qua non* per dare solidità al pluralismo culturale e dell'informazione, senza i quali la stessa democrazia rischia di essere svuotata di significato. Questo era il senso il senso del disegno di legge Gentiloni che abbiamo cercato di far approvare nella scorsa legislatura, purtroppo terminata anticipatamente. Chiediamo, inoltre, che il Parlamento, attraverso le Commissioni competenti, venga permanentemente informato del programma di digitalizzazione che certamente deve avere nell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e nel Ministero competente la responsabilità di programmazione e di attuazione.

Ciò significherebbe dare carta bianca ad un Governo che, come si vede, ha costantemente bisogno dell'attenzione vigile dell'opposizione, e ad una maggioranza che in questi ultimi due anni,

Guardiamo però al primo atto del governo Berlusconi in materia: il taglio dei 50 milioni di euro del fondo per lo sviluppo della banda larga e dei 20 milioni di euro del fondo per il passaggio al digitale terrestre, tagliati insieme a tanti altri provvedimenti per finanziare lo sgravio fiscale dell'ICI e degli straordinari. Questi sono gli atti concreti del Governo, che rispondono bene al senatore Butti. Consentitemi, infine, di illustrare

per i prossimi 30 anni la concessionaria del gruppo Benetton si è assicurata aumenti tariffari garantiti, con un flusso di cassa stimato al 2038 a quasi due miliardi. Lo Stato, inoltre, rinuncia di fatto ai controlli sui costi. Come è noto, ciò è dovuto al riconoscimento ad ASPI di una formula tariffaria innovativa e molto, molto preferenziale; qualcuno ha sospettato, in questa Aula e anche alla Camera, che questa preferenza sia connessa alla cordata (per il momento fantasma) relativa ad Alitalia. Si è reintrodotta in questo modo una sorta di scala mobile, abolita più di 20 anni fa; ma la si è reintrodotta non per i pensionati, come promesso dal PdL in campagna elettorale, ma per i quasi monopolisti proprietari di ASPI. È una scala mobile che sarà pagata dai pendolari e che inciderà sull'inflazione! Il ministro Tremonti minaccia una Robin Hood *tax*: questo è il primo esempio di un intervento, che è però Robin Hood alla rovescia! Per queste ragioni,

risentono, ovviamente, del periodo di transizione tra un Governo e l'altro. Come sempre accade, si intrecciano valutazioni contrapposte

né da vituperare particolarmente. È un provvedimento elaborato dal Governo precedente e che voi, colleghi dell'opposizione, faticate a ripudiare come figlio del vostro Governo; nello stesso tempo, si tratta di un provvedimento con margini molto necessitati. Si è trattato, in buona sostanza, di un testo che ha dovuto venire incontro ad esigenze oggettive di urgenza,

che vanno dalla discriminazione delle persone in ragione delle loro qualità e delle attività svolte, alla protezione delle vittime, a tutto il caldo tema delle frequenze radiotelevisive,

mi permetterete di non ritornare sui singoli passi che sono stati oggetto degli interventi tematici degli onorevoli colleghi e che hanno trovato delle risposte - mi sembra - abbastanza satisfattive e concludenti da parte sia del Sottosegretario, onorevole Romani, che del relatore, senatore Malan. Quando però un'opposizione vuole presentare metà volto dialogante

vi siete dibattuti nella grande difficoltà di dover votare contro per voler evidenziare un vostro ruolo di opposizione rispetto a presunti sconvolgimenti che la nuova maggioranza avrebbe apportato al testo, e di non negare le esigenze che avevano spinto il vostro - e non il nostro - Governo a predisporre questo testo. Comprendiamo le vostre difficoltà. Non vi lanciamo contro naturalmente respingiamo qualche anatema e qualche tono troppo emotivo ed enfatizzato a cui taluni degli oratori dell'opposizione si sono abbandonati. In realtà, noi, come Gruppo di maggioranza, in sintonia con il nostro Governo, esprimeremo voto favorevole - complessivamente parlando - per quel senso di responsabilità che un Governo subentrante e la sua maggioranza debbono manifestare. D'altronde, sui punti più delicati o che sembravano tali, i chiarimenti sono stati forniti, non dico a questo punto a chi non li vuole ascoltare o a chi non li vuole capire, ma soprattutto al Paese, all'opinione pubblica che resta il nostro sovrano interlocutore. Del resto, la norma più controversa a volerla considerare tale - che era appunto quella riguardante la materia radiotelevisiva, non per nulla è stata sottratta, è sfilata via dal dibattito. In sede di Camera dei deputati è stata così incisivamente ritirata e comunque si sarebbe dovuto supporre che avesse dato luogo ad una pronuncia di cessata materia del contendere; ma chi vuole mantenere alto il livello della contesa evidentemente a questo non si rassegna. Le altre norme non sono tutte degne di un dieci e lode. Non abbiamo nessuna difficoltà a darne atto, perché ci si è dovuti muovere in un terreno già arato, in una situazione di emergenza, attraverso una pronuncia della Corte costituzionale che - come hanno detto diversi di voi - non risolve tutti i problemi; apre la strada a soluzioni, incoraggia, stimola, indica delle strade di soluzione ma - anche perché non è suo compito - non tutte le risolve né permette di considerarle esaurite. Abbiamo quindi dovuto tenere conto - tutti dovremmo tenere conto - di questo tipo di pronunce. sono motivazioni di sintesi di valutazione politica che credo non possiate accusare di faziosità o di partito preso: rappresentano l'equilibrio tra le esigenze che ci vengono da scelte di carattere nazionale - sulle quali rivendichiamo il diritto non solo del precedente Governo, ma certamente anche di questo di tutelare la volontà di scelta del governo sovrano della nostra Nazione - e quello di essere leali e rigorosi e non più inadempienti. Tutti, infatti, riconosciamo che dobbiamo recuperare molto terreno e risalire la china delle infrazioni e delle inadempienze rispetto alla Comunità europea. Sulla base di questa cultura di Governo, di queste valutazioni che credo siano un ragionevole punto di equilibrio tra diverse esigenze, molte delle quali non da noi create, riteniamo giusto giusto allungare il passo in questa fase di transizione tra un Governo e l'altro, rimandando a provvedimenti - l'ha detto il Governo stesso - che non mancheranno di venire per riempire i vuoti

Come molti ricorderanno, all'articolo 1, comma 376, di quella finanziaria, si stabilì

1999. Si aggiunse anche la norma secondo la quale il numero complessivo dei Ministri, dei Vice ministri e dei Sottosegretari non poteva essere superiore a 60. Al successivo comma 377 vennero abrogate una serie di disposizioni incompatibili con il comma precedente e si fecero invece espressamente salve alcune norme. norme. Il Governo Berlusconi si è adeguato completamente a questa normativa ed è intervenuto richiamandosi al decreto legislativo n. 300 del 1999, indicato con il nome di Bassanini, per avere esattamente lo stesso organico di quel testo legislativo. Sappiamo che questa situazione di adeguamento non era necessaria sul piano normativo, in quanto quella disposizione della legge finanziaria 2008 aveva lo stesso rango dell'attuale provvedimento d'urgenza.

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero per i beni e le attività culturali. Rispetto all'imperio della finanziaria, secondo cui bisognava rispettare soltanto il numero dei Ministeri indicati nel vecchio decreto legislativo

Ecco quindi che si spiega questo provvedimento che nella prima parte vede la normazione ho ricordato. Esso introduce poi una serie di adeguamenti con vari trasferimenti, una massiccia attribuzione di materie alla Presidenza del Consiglio, la necessità espressa di risparmiare a fine percorso, dopo i processi di riallocazione e mobilità del personale, almeno il 20

e oggettivo per lo Stato. Norme diverse sono soltanto quelle di cui al comma 21,

un Ministro o un Sottosegretario dell'attuale Governo possa assumereanche la funzione di autorità delegata, ai sensi della legge sui Un'ultima notazione riguarda il processo di scelta di magistrati e altri funzionari per la collocazione alle dipendenze dei Ministri. Dopo le parole

illustrato le caratteristiche generali del disegno di legge di conversione del decreto riguardante la struttura del Governo, che abbiamo peraltro esaminato in Commissione affari costituzionali. Ci troviamo di fronte all'attuazione di una norma significativa, poiché tutti ricordiamo nella scorsa legislatura quanto l'opinione pubblica sia stata coinvolta

La struttura del Governo ed il numero dei Ministeri costituiscono aspetti fondamentali

Il primo è che è necessario rendere più snella la compagine di Governo, riducendo il numero dei Ministri, dei Vice ministri e dei Sottosegretari. La norma approvata con la finanziaria 2008, ricordata dal collega Boscetto, prevede che i componenti a qualunque titolo del Governo non possano superare le 60 unità.

Con la norma della legge finanziaria 2008 si prevede di tornare esattamente a quella disposizione. I Ministeri debbono essere 12 e il numero dei componenti complessivi del Governo non può eccedere le 60 unità. Il decreto che ci viene sottoposto recepisce la norma della finanziaria

In Commissione ne abbiamo ragionato ed è venuta dal Governo e dalla maggioranza anche una certa disponibilità ad esaminare successivamente il problema. Resta comunque ferma la necessità di ottemperare a quanto dispone la finanziaria per il 2008 per quanto riguarda la riduzione del numero dei Ministeri. anche un problema di efficienza della macchina amministrativa, perché non c'è dubbio che aver diviso certi Ministeri, com'è avvenuto, ripeto, in entrambe le legislature precedenti, rispetto all'ipotesi originaria del decreto legislativo n. 300, ha reso più farraginosa e difficile l'azione di Governo. Anche la frantumazione politica e l'estrema eterogeneità delle coalizioni, che hanno caratterizzato in modo particolare la legislatura precedente, hanno inciso molto sulla composizione del Governo dal punto di vista della sua pletoricità. Tutti i Governi che si sono succeduti nelle ultime due legislature hanno sicuramente sofferto di questo problema. Il decreto comporta il trasferimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili e di politiche per la famiglia. Il Centro nazionale documentazione ed analisi per l'infanzia e l'adolescenza viene trasferito alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Vi è, inoltre, la norma che ricordava il collega Boscetto, relativa al fatto che il membro di Governo che ha la delega per i Servizi di informazione e sicurezza può avere anche altre deleghe, in deroga alla riforma dei Servizi che, peraltro, è stata approvata all'unanimità nella scorsa legislatura. Per il resto, ripeto, il decreto

In Commissione, oltre all'emendamento di cui ho parlato relativo al Ministero della salute, abbiamo esaminato un emendamento da me presentato me presentato che si riferisce alla necessità di introdurre un Coordinamento interministeriale per le politiche urbane, di cui parleremo naturalmente nel corso della discussione. In modo particolare, da parte nostra è stata sollevata una questione rispetto alla quale, in Commissione, sia il relatore che il Governo hanno mostrato sensibilità.

Però, evidentemente, l'Esecutivo si è reso conto che non si poteva derogare così semplicemente e lo ha fatto con parole che dimostrano l'eccezionalità di quel provvedimento. Infatti, nel decreto sull'emergenza rifiuti in Campania via di assoluta irripetibilità e straordinarietà per far fronte alla gravissima situazione in corso e comunque fino al 31 dicembre 2009». Queste sono le parole, il contenuto della norma si riferisce all'introduzione della figura del Sottosegretario presso la Presidenza del Consiglio che è delegato, appunto, alla protezione civile e, in modo particolare, all'emergenza rifiuti in Campania. I componenti del Ora, noi siamo preoccupati per alcune dichiarazioni che abbiamo letto sulla stampa, rese sia da autorevolissimi esponenti del Governo che da esponenti della maggioranza, in base alle quali ci sarebbe l'intenzione, tra qualche mese, di proporre provvedimenti che allargano il numero dei componenti del Governo, magari introducendo la figura dei Vice ministri. Sia chiaro, signori rappresentanti della maggioranza e signori del Governo,

ci fosse l'intenzione di presentarvi nelle Aule del Parlamento per proporre un allargamento della compagine di Governo, avreste la nostra più piena e totale contrarietà

Non ci sono ragioni di operatività che richiedano un aumento del numero dei suoi componenti. annuncio che il nostro Gruppo presenterà, in sostituzione di uno degli emendamenti, un ordine del giorno che abbiamo già discusso in Commissione con il quale impegniamo il Governo a non proporre altre deroghe al numero totale dei componenti,

che «la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini» ai fini dell'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive. Riteniamo che

anche se ci sono state illustrate le ragioni del provvedimento. Sicuramente non è stato bene modificare una legge, che aveva una propria collocazione, in una sede come questa e, soprattutto, forse non è stato bene aver abrogato aver abrogato un articolo che aveva una propria *ratio*, quella cioè che l'Autorità delegata dal Presidente del Consiglio per i Servizi di sicurezza fosse esonerata da qualsiasi altro incarico.

oggi, con il disegno di legge di conversione, si provvede al riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri attraverso quanto già previsto dall'articolo 1, commi 376 e 377,

vengono trasferite al Ministero dello sviluppo economico le competenze e le relative risorse attribuite nel precedente assetto organizzativo al Ministero del commercio internazionale. Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie e strumentali, le funzioni attribuite al Ministero dei trasporti. Per quanto concerne le competenze del soppresso Ministero della solidarietà sociale, il decreto disciplina il trasferimento di alcune funzioni, con le inerenti risorse finanziarie e strumentali, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e attribuisce nuovamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con le inerenti risorse, funzioni prima spettanti al Ministero della solidarietà sociale.

Con riferimento, in particolare, all'ordinamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, va ricordato come l'Italia dei Valori abbia espresso alcune riserve sul cosiddetto spacchettamento dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti che fu necessario operare nella scorsa legislatura, attraverso il decreto-legge n. 181 del 2006. quindi dirsi contraria, in linea generale, al ritorno dell'articolo 55 del decreto legislativo n. 300 del 1999, che disponeva la nascita del Ministero unificato, accorpando le funzioni ed i compiti del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dei trasporti e della navigazione, nonché del Dipartimento per le aree urbane istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Tuttavia va anche ricordato che nella scorsa legislatura, pur nello spazio temporale concesso dalla sua breve durata, si è avviato un positivo processo di razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi dei Ministeri, e del Ministero delle infrastrutture in particolare, attraverso l'emanazione di specifici regolamenti, secondo un programma di riorganizzazione, previsto dal comma 404 dell'articolo 1 della finanziaria 2007, finalizzato appunto al contenimento delle spese di funzionamento. Si tratta di un processo che auspichiamo sia salvaguardato, al di là dei risparmi di spesa che sono attesi dall'unificazione dei due Ministeri.

Innanzitutto, sotto il profilo del *drafting* redazionale, il decreto accorpa sotto l'unico articolo 1 ben 24 commi di differente contenuto normativo: la ridefinizione dei Ministeri, la loro riorganizzazione amministrativa, le nuove denominazioni, nonché l'abrogazione di un comma di una norma ordinamentale assai rilevante, quale quella della riforma dei Servizi. Si propone, dunque, l'inserimento di più articoli con le rispettive rubriche. Inoltre, nell'ottica di una riorganizzazione razionale ed efficiente della struttura di Governo, pur risultando assai apprezzabile lo snellimento delle strutture ministeriali, si rileva come l'accorpamento del Ministero della salute nel Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali possa risultare assai problematico. Nel nostro ordinamento non vi sarà o sarò molto difficile avere un coordinamento centrale ed una figura di riferimento autorevole per i problemi dei pazienti e del personale sanitario. È chiaro, infatti, che il Ministro del *welfare*, unico a sedersi in Consiglio dei ministri, si preoccuperà dell'equilibrio finanziario complessivo della sanità e, contestualmente, di quello degli altri fondamentali settori che egli rappresenta: politiche sociali e del lavoro. Nonostante tali funzioni vengano giuridicamente assunte da un Sottosegretario, sotto il profilo politico è soltanto con la presenza di un Ministro che si riconosce ad un particolare settore un'importanza strategica e cruciale per la vita dei cittadini e per la loro sicurezza sociale. Si ricorda, a questo proposito, che l'articolo 32 della nostra Costituzione indica che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. Si sottolinea, infine, che anche nella prospettiva dell'introduzione del federalismo fiscale appare assolutamente necessario un riferimento nazionale, "guardiano" dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale. rilevato che l'accorpamento dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti dovrà essere operato evitando sovrapposizioni interne e problemi alla efficacia e funzionalità delle strutture, ma in particolare valorizzando l'opera positiva di riorganizzazione che, come ho già detto, ha conosciuto il Ministero delle infrastrutture nei due anni trascorsi. Il regolamento di riorganizzazione di tale Ministero è già stato adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2007, ridisciplinando l'esercizio delle funzioni di programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti infrastrutturali di interesse nazionale, ivi comprese le reti elettriche, idrauliche e acquedottistiche, e delle altre opere pubbliche di competenza dello Stato; la qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; le costruzioni nelle zone sismiche; l'edilizia residenziale e le politiche dell'edilizia concernenti anche il sistema delle città e delle aree metropolitane; sicurezza e la regolazione tecnica, e così via. Il regolamento di riorganizzazione del Ministero riguarda non solo le 11 direzioni generali, ma anche il Consiglio superiore dei lavori pubblici e gli incarichi di livello dirigenziale generale con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca. L'accorpamento dovrebbe quindi salvaguardare le positive innovazioni conosciute dalla struttura nel periodo 2006-2008 e consolidare i risultati raggiunti. Ancora. La drastica riduzione del numero dei Sottosegretari di Stato potrebbe determinare un rallentamento dei lavori parlamentari in Aula, oltre che in Commissione. ultimo, la legge finanziaria 2008, nei commi sui cui tale decreto incide, ribadisce un fondamentale principio costituzionale: la composizione del Governo dovrà essere configurata «in coerenza» con il principio di cui all'articolo 51, primo comma, secondo periodo, della Costituzione, secondo cui la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini ai fini dell'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive. Rileviamo come l'attuale composizione governativa non corrisponda esattamente a detti princìpi, valutata la assoluta minoranza del genere femminile sia tra i Ministri che tra i Sottosegretari di Stato.

Signora Presidente, onorevoli senatrici e senatori, nel proporre con un emendamento l'istituzione del Ministero della salute avrei l'obiettivo di colmare una grave e a mio avviso pericolosa mancanza nell'attuale organizzazione del Governo del nostro Paese. Non istituendo il Ministero della salute, per la prima volta nella storia dell'Italia, si è determinato un vuoto ai vertici della sanità nazionale. Certo, possiamo vantarci di essere stati i primi in Europa e forse anche nel mondo ad aver fatto questa scelta, ma permettetemi di dire che si tratta di una scelta anomala e sbagliata, che causerà gravi problemi e disfunzioni al corretto funzionamento del Servizio sanitario nazionale. La decisione non è stata di tipo tecnico, come alcuni sostengono. Come sappiamo bene, infatti, la legge finanziaria per il 2008 ha ripristinato solo il numero dei Ministeri, riflettendo quanto già previsto nel 1999, ma non anche non anche l'originaria denominazione e la ripartizione delle attribuzione fra di essi. Per essere più chiari, la legge non indica espressamente quali Ministeri devono essere soppressi rispetto a quelli che esistevano nel precedente Governo e non indica quali devono esercitarne le competenze. La legge indica semplicemente che i Ministeri devono essere 12, ma lascia la libertà di indicare quali sopprimere e quali mantenere. In questo senso, non si può negare che l'abolizione del Ministero della salute sia stato il frutto di una decisione politica e che tale decisione possa trasmettere a medici, infermieri e a tutti i cittadini del nostro Paese il messaggio di uno scarso interesse, da parte delle forze politiche di centrodestra, verso la tutela dei dritti e della salute dei cittadini italiani. Se infatti spetta alle Regioni amministrare la quotidianità dei servizi sanitari, gestire le strutture, gli ospedali, organizzare tutti i servizi sanitari sul territorio, è compito però del Governo centrale fare sì che questi servizi siano garantiti in maniera corretta ed omogenea su tutto il territorio nazionale. Questo non accade, lo sappiamo bene, ma senza una guida, senza un'azione di coordinamento e di controllo a livello centrale, senza una figura autorevole come quella di un Ministro, il principio dell'uguaglianza e dell'omogeneità sarà messo in discussione ancora di più. E alcuni cittadini saranno ancora una volta vittime di questa discriminazione. Un Governo che si vuole garante di tutti i cittadini non può ignorare gli enormi problemi delle Regioni del Sud, soprattutto in sanità, e lasciare che il divario tra le Regioni diventi ancora più ampio e che questo ricada sulla salute dei cittadini. Serve un coordinamento centrale forte, serve un punto di riferimento che si occupi di guidare la sanità, di monitorare i servizi, di valutare carenze e mancanze dove esistono e non semplicemente di assistere alle scelte fatte a livello regionale. Senza questo ruolo importantissimo di guida il Servizio sanitario nazionale sarà inevitabilmente indebolito a favore di 20 sistemi diversi, alcuni buoni, altri purtroppo meno buoni. Inoltre, la presenza di un Ministro della salute è fondamentale per permettere all'Italia di far sentire la propria voce in ambito internazionale quando i vertici dei Paesi europei ed extraeuropei si troveranno a discutere delle tante emergenze sanitarie che riguardano l'intero pianeta. Per tutti questi motivi, faccio appello al senso di responsabilità di quest'Aula affinché esprima voto favorevole all'emendamento che ripristina il Ministero della salute. Sono certo che molti membri della maggioranza con cui ho lavorato anche nella passata legislatura condividono le mie preoccupazioni e mi auguro che con il contributo di tutti si possa porre rimedio alla situazione attuale, riconoscendo che la cancellazione del Ministero è stata un errore e che per correggerlo è sufficiente il voto positivo dell'Aula. *(Applausi

di una pessima abitudine perché l'utilizzazione del decreto-legge comporta la scomposizione e ricomposizione di Ministeri, dipartimenti e quant'altro, vulnerando uno dei principi fondamentali su cui si regge l'attività amministrativa, vale a dire il principio della continuità. Poiché la passata legislatura, come è noto, è durata solo due anni,

Da questo punto di vista riteniamo che il provvedimento presentato dal Governo abbia queste caratteristiche. Certo, credo che la via maestra sarebbe quella di lavorare sulla riforma della Presidenza del Consiglio e, anziché utilizzare il decreto-legge, intervenire sulla legge n.

normativi secondari, riorganizzare o riaccorpare le funzioni amministrative e ministeriali in ragione delle priorità dell'azione di Governo individuata. Tutto questo consentirebbe anche di non vulnerare il principio della continuità amministrativa che credo sia estremamente importante.

Proprio questa nuova riorganizzazione ha determinato la valutazione unanime del Parlamento di evitare che il Ministro o il Sottosegretario delegato a seguire i Servizi potesse occuparsi anche di altri settori. Pertanto, per la verità, a noi qualche dubbio, con riferimento all'operatività della riforma, lo pone la soppressione dell'esclusività dei compiti e delle funzioni dell'Autorità delegata, delegata, anche riguardo al rafforzamento dei poteri di controllo e di decisione che in questa materia la legge di riforma ha attribuito al Parlamento. Quindi, la necessità di avere un'autorità politica, che poi ha rilevanti compiti non solo di responsabilità politica ma anche operativi in questo settore, che deve lavorare a stretto contatto con il Copasir, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, ci aveva portato a fare questo tipo di valutazione. Comprendiamo che è è anche necessario tenere conto di fatti e di esigenze particolari e quindi è anche corretto che in qualche modo si possa intervenire; intervenire; non abbiamo presentato emendamenti su tale aspetto e non ne presenteremo; non ne abbiamo presentati per nessuna delle questioni che sono disciplinate dal decreto-legge, ma in modo particolare su questo punto - ripeto - sottolineiamo questa perplessità perché non riusciamo a comprendere quale sia la logica sottesa all'abrogazione di questa norma fondamentale, dal nostro punto di vista, per l'attuazione di una riforma così importante che è venuta dopo trent'anni dalla precedente legge che ha disciplinato i servizi di *intelligence* nel nostro Paese. L'ultima considerazione

a venire incontro a tale esigenza - nella fase transitoria (una fase abbastanza lunga di risistemazione e riorganizzazione dei singoli Ministeri con lo spacchettamento di alcune deleghe e di alcuni settori e la ricomposizione in altri

complessiva, un'attenzione in più e particolare al regime transitorio anche in via di attuazione, con normative di carattere regolamentare che consentano sostanzialmente di non paralizzare o di non bloccare alcuni settori strategici. Mi riferisco, ad esempio, allo sviluppo economico, ma questo riguarda anche la nuova riorganizzazione e la rinascita del *welfare*, del sistema del *welfare* complessivamente considerato; questa attività di riorganizzazione non paralizzare l'azione e l'attività amministrativa perché credo che ne deriverebbero dei problemi in più. Già di problemi ne abbiamo tanti; se qualcuno riusciamo a risparmiarcelo non sarebbe male. Queste sono le ragioni per le quali anticipiamo il nostro voto di astensione

Signora Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli senatrici e senatori, mi soffermerò brevemente soltanto sul comma 4 dell'articolo 1, anche perché mi sembra siano state le osservazioni dominanti fino a questo momento in Aula. Nel passaggio del decreto-legge in esame nella Commissione igiene e sanità vi è stato un coro unanime, racchiuso tra l'altro in una dichiarazione finale votata all'unanimità, in cui si sottolineava al Governo una raccomandazione, ossia che possa tornare a vivere il Ministero della salute; possa ritornare a vivere soprattutto in un momento di attenzione non negativa da nessuna parte dello Stato o della Nazione nei confronti del federalismo fiscale. Anzi, onde accentuarne caratteristiche solidali, tra l'altro così richiamate anche dal Presidente della Repubblica, l'intera Commissione si esprimeva raccomandando che tornasse un momento di attenzione unitaria nella gestione, nella programmazione, nell'attenzione socio-sanitaria, nei confronti di qualsiasi latitudine o longitudine, di qualsiasi ceto sociale. È più facile ritrovare questi motivi di garanzia in un Ministero *ad hoc* deputato, anche se non è qualcosa che vorremmo che si verificasse in questo momento. Certamente, comprendiamo le attenzioni circa il rispetto nei confronti della finanziaria del 2008 e dell'applicazione del decreto legislativo n. Riteniamo, però, che questa attenzione possa determinare momenti di risposta concreta alle aspettative di tutte le popolazioni che intendono avere qualità, quantità, innovazione tecnologica, attenzione e certezza di percorsi nella risposta ai bisogni della salute. Questa è una sensibilità che, in modo ingeneroso probabilmente, il senatore Marino non riconosceva al centrodestra. Voglio ricordare che il Governo Berlusconi nel 2001 ha voluto il Ministero della salute. Quindi, è un'attenzione concreta che si può esprimere anche nell'attuale legislatura e che può trovare una risposta adeguata a queste esigenze e anche ad una rappresentazione plastica dell'attenzione dello Stato nei confronti di esigenze primarie e comuni. Oggi, nella sanità

delle amministrazioni regionali di esprimersi sempre con la visione del bene comune: molto spesso vi sono deviazioni dai concetti di sicurezza per la tutela della salute.

con una conseguente redistribuzione di competenze e deleghe; per questo motivo, ritengo sia forte il consenso per la conversione in legge di un decreto-legge che riguarda una materia rispetto alla quale la sensibilità dei cittadini è altissima. Ho sentito dire che lo strumento del decreto-legge per la riorganizzazione della struttura di Governo è il meno indicato. A mio giudizio, un Governo che entra in carica che vince le elezioni ha tutto il diritto di adottare uno strumento immediato per poter dare attuazione al programma presentato agli elettori e per creare il suo Esecutivo, in maniera tale che questo possa operare nell'immediatezza.

la programmazione di un Esecutivo preposto a risolvere i problemi del Paese. Voglio qui ricordare che in questa

il centrosinistra, che stasera fa certe affermazioni, aveva speso ricette ed etica a buon mercato per dire che bisognava moralizzare la vita pubblica a cominciare dalle auto blu; ricordo bene quelle dichiarazioni. Certo, è stato difficile tagliare le gomme al parco macchine se poi dagli allora Ministri in giù si era dato vita un corteo infinito di cariche, che a loro volta moltiplicavano le sotto cariche e gli incarichi. Ma questa ormai è acqua passata. Si è voltata pagina e siamo in presenza di una nuova mappa di Governo, frutto di una analisi e di un censimento dettagliato delle esigenze di affidare deleghe e competenze in modo specifico e settoriale ma con razionalità, efficacia ed efficienza - dico io - perché sappiamo bene che una eccessiva parcellizzazione delle competenze genera conflitti. È È stata osservata - l'abbiamo già ricordato - una linea base stabilita dalla finanziaria del 2008 e non solo. Ha ricordato bene oggi il senatore Boscetto, in sede di 1a Commissione, che i Ministeri sono quelli definiti dalla riforma Bassanini, almeno per quanto riguarda i primi 12. Ho già detto che si può voltare pagina e scrivere un lustro di storia nazionale caratterizzata dalle riforme, da un profondo cambiamento della società italiana. È una sfida ha tante difficoltà legate alla congiuntura economica internazionale, a tutte quelle incrostazioni che hanno incancrenito i problemi, i disagi e le ingiustizie sociali. L'accento è stato posto in modo particolare sulla mancata previsione di un Ministero *ad hoc* per la sanità. non si può parlare di discriminazione di cittadini che non sono tutelati perché manca un Ministero specifico per quella materia. È una materia prevista nell'ambito di un altro Ministero. È stato detto che occorre anche un periodo di rodaggio per vedere come le situazioni si svilupperanno e si modificheranno, se ce ne sarà la necessità. lo spazio è ampio per dire tutto e il contrario di tutto: ad esempio anche il Ministero dell'ambiente - se vogliamo - potrebbe essere accorpato al Ministero dell'industria piuttosto che a quello delle infrastrutture, perché l'ambiente tratta tutte le problematiche inerenti alle attività umane, alle infrastrutture, alla costruzione di grandi opere per fare una valutazione di impatto ambientale, all'emissione in atmosfera di tutte le attività produttive e via dicendo. certamente affermare di tutto e di più, ma questo non vuole dire che non prevedere certe cose discrimini i cittadini italiani. Quindi, in linea generale e arrivando anche alla conclusione, esprimiamo

proponendo una compagine governativa snella e ben strutturata e in linea con le previsioni dell'ultima finanziaria del Governo Prodi e della riforma Bassanini. Il radicale ripensamento dell'organizzazione ministeriale appare una conquista importante non solo sul piano politico ma anche su quello più propriamente finanziario ed organizzativo. È importante evidenziare anche questo aspetto, ossia il piano finanziario: la razionalizzazione delle cariche di Governo si pone perfettamente in linea con il tema della riduzione dei costi della politica, che non solo ha rappresentato il *leitmotiv* dell'ultima campagna elettorale ma soprattutto si impone come primario obiettivo di Governo al fine di superare quella disaffezione degli elettori nei confronti della politica, emersa chiaramente nel dibattito politico e mediatico degli ultimi mesi. In conclusione, vorrei esprimere esprimere l'augurio che dalla presente riorganizzazione possa derivare un'azione di Governo realmente innovativa nella sua efficacia e nella sua effettività. Penso che già dalle prime settimane, ministro Vito, il Governo abbia dimostrato di operare con determinazione e incisività. Nel medio e lungo periodo è auspicabile che la ristrutturazione del Governo possa possa estendersi anche ad una riforma complessiva del Parlamento, finalizzata, in particolare, alla riduzione del numero dei parlamentari e alla trasformazione del Senato in un'Assemblea di stampo federalista.

«E chiederemo politiche sociali audaci e impegnative. Il nostro è un grande sì alla famiglia che, siamo certi, incontra la ragione e il cuore degli italiani». Senza dubbio molti di noi condividono queste parole, al di là dei diversi approcci alla famiglia. L'abolizione del Ministero della famiglia e la sottrazione delle deleghe ad altri Ministeri competenti, previste dal presente decreto, rispondono alle richieste del manifesto di politiche sociali audaci e impegnative? Incontra la ragione e il cuore degli italiani l'aver delegato tutto ad un sottosegretario presso la Presidenza del Consiglio? Per rispondere a queste domande occorre richiamare alcune delle motivazioni che portarono il centrosinistra ad istituire il Ministero della famiglia e ad indire la prima Conferenza della famiglia a Firenze nel 2007, alla presenza dello stesso presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. La prima ragione della scelta di istituire il Ministero della famiglia va ricercata nella crescente consapevolezza e nella stessa umiltà con cui si è preso atto dell'enorme ritardo con cui il nostro Paese ha affrontato i grandi cambiamenti che sono intervenuti nelle famiglie. La vita delle famiglie in pochi decenni è cambiata in misura maggiore di quanto abbia fatto negli ultimi due secoli. Non c'è ambito della vita nazionale, così come, con la globalizzazione, nella vita internazionale, che non produca sollecitazioni nuove nella vita familiare: dal numero dei componenti delle famiglie, alla vita media, al tipo di famiglia, ai rapporti tra i generi e le generazioni, ogni aspetto è cambiato. Molti Paesi europei, in questi decenni, pur partendo da posizioni più avanzate delle nostre, hanno rivisto le proprie politiche relative a investimenti, strumenti e legislazioni. In Italia, nonostante leggi importanti, non siamo ancora riusciti a sviluppare forti e adeguate politiche pubbliche. La stessa legge n. 328 del 2000, incrociando la riforma del Titolo V, e priva della scrittura dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, non ha potuto sviluppare per intero il suo potenziale. Per tale motivo, alla conferenza di Firenze, il ministro Bindi ha proposto i livelli essenziali per la famiglia, anche per incidere sull'enorme divario tra Nord e Sud: ad esempio, la povertà delle famiglie al Sud è cinque volte più elevata che al Nord. Il Ministero della famiglia è nato proprio per far compiere un balzo in avanti nel sostegno alla famiglia. La seconda ragione consiste nel ritenere indispensabile un luogo pubblico autorevole e riconosciuto in cui mettere al centro la famiglia rifuggendo da qualsiasi familismo che ha reso più fragile, solo e non riconosciuto ogni componente della famiglia. La famiglia è risorsa e le politiche pubbliche hanno senso e forza solo se riconoscono tale principio; ma la famiglia è risorsa se non è lasciata sola, se è messa in grado di essere protagonista e se ha tutti gli aiuti necessari per affrontare il proprio quotidiano e i momenti in cui nella vita conosce maggiori difficoltà. Il familismo è l'esatto contrario del riconoscimento del valore della famiglia. Il familismo, dietro la sua retorica, nasconde la solitudine della famiglia e l'indifferenza dello Stato. È l'opposto di politiche pubbliche moderne a sostegno delle famiglie e ci imprigiona in ciò che gli studiosi chiamano *welfare* mediterraneo, di cui l'Italia, spendendo meno della metà della media europea per le famiglie e dedicando ancor meno risorse ai servizi, è una rappresentante significativa. Il risultato è una famiglia sempre più piccola e anziana. La sua costituzione slitta di più nel tempo, fa pochi figli, che rimangono a casa molto più a lungo dei propri coetanei d'Europa. Le donne che lavorano sono poche e lo fanno con enorme difficoltà per l'impossibilità di conciliare i tempi del lavoro e degli affetti. Per questo penso che ognuno di noi sia toccato dalla tragedia di Simona Verzelletti. Per questo riteniamo un errore abolire il Ministero. In questi anni il Paese sa che è importante la sua unità su temi così delicati. La stessa Conferenza di Firenze aveva fatto fare dei passi in avanti, in particolare su due aspetti fondamentali: il riconoscimento sia dei diritti della famiglia che dei diritti inviolabili della persona e il legame, strettissimo, tra promozione della famiglia e crescita del Paese. Un grande Paese sa che è tale perché è capace di guardare oltre l'oggi: quindi, di investire sapendo che se i costi sono immediati i benefici sono distribuiti sull'intero arco della vita. Nell'economia della conoscenza il più lungimirante investimento sul capitale umano è quello sui bambini. La formazione e l'educazione fin dai nidi sono la leva decisiva per ridisegnare le politiche contro le disuguaglianze, condividere il progetto educativo e rendere il Paese competitivo. Le famiglie da sole non possono farcela, questo è un compito che riguarda l'intero Paese.

è la terza legislatura consecutiva che si apre con un provvedimento urgente in materia di struttura del Governo, di numero dei Ministeri, di funzioni dell'Esecutivo. Le motivazioni di questi tre decreti-legge sono state diverse, ma tutte e tre hanno oggettivamente determinato e determinano oggi un momento di difficoltà perché ristrutturare l'organizzazione ministeriale significa intervenire su funzioni, risorse, uomini e beni di varia natura senza i quali o a dispetto dei quali non si può portare avanti nessuna azione concreta. Il primo decreto-legge che voglio ricordare è quello che adottò il Governo Berlusconi nel 2001, ma ricordiamoci pure che quel decreto-legge fu reso necessario da una riforma, introdotta con il decreto legislativo n. 300 del 1999, che veramente rivoluzionò il sistema dell'organizzazione del Governo. La riforma Bassanini intervenne in maniera radicale portando a 12 i Ministeri, realizzando degli accorpamenti certamente discutibili,

quindi, materie che si riteneva avessero un minore impatto sull'attività del Governo nazionale. Così poi non è stato e pertanto il Governo Berlusconi nel 2001, nell'affrontare la prima esperienza di quel quinquennio di continuità governativa, ritenne di spacchettare due Ministeri, che poi oggi vengono invocati anche da tanti dell'opposizione, vale a dire il Ministero della salute e quello delle comunicazioni. E lì si fermò

ha messo nel cassetto la riforma Bassanini (strano destino per una riforma approvata dal centrosinistra e poi annichilita, rovesciata, travolta da un Governo di centrosinistra):

e credo che non poco abbia pesato quella fase di riorganizzazione sull'inefficienza universalmente riconosciuta di quel Governo.

positivamente, in quanto, considerando gli uffici pubblici come uffici di servizio per i cittadini e non come mezzi esclusivamente destinati a soddisfare le esigenze e gli equilibri politici più o meno legittimi,

componenti in totale, compresi i Ministri, i Vice ministri ed i Sottosegretari che non siano Vice ministri. Ritengo che allora c'era una ventata di antipolitica, anche giustificata - forse c'è ancora adesso - che portava a radicalizzare certe scelte legislative. Oggi mi fa piacere che il Governo con questo decreto‑legge sostanzialmente onori nella forma, oltre che nella sostanza, quanto stabilito dalla finanziaria, ripristinando il numero dei Ministeri previsti, senza creare quelle disfunzioni che invece le riforme precedenti, dapprima la Bassanini e poi quella di Prodi, avevano determinato. Certamente, anche per questo Governo vi sarà la necessità di passare questo guado per arrivare ad una ristrutturazione definitiva della compagine governativa. Bisognerà allora anche chiedersi

Mi rendo perfettamente conto - ciò è avvenuto e qui dobbiamo testimoniarlo - che ogni Commissione ha al di là dello schieramento dell'uno o dell'altro collega senatore, la necessità che emergesse la particolarità e la rilevanza di un certo settore, soprattutto se oggi strutturato nei megaministeri che abbiamo dinanzi

ai colleghi che hanno assunto ad esempio la mancata previsione del Ministero della salute come Ministero a sé stante, posta la necessità di mantenere in

l'opposizione, che oggettivamente non manca occasione per contestarci scelte che possono apparire, e magari sono, impopolari. Un'altra osservazione, Presidente, e mi avvio a concludere, sulla questione relativa alla modifica della legge di riforma dei Servizi segreti.

Sono stato relatore di tale provvedimento in Senato ed è stato questo un punto del quale si è discusso, soprattutto nell'ambito di una ristrutturazione dei Servizi che ha incardinato in capo al Presidente del Consiglio dei ministri le responsabilità della gestione e delle azioni dei servizi di *intelligence*. Questa è la novità maggiore oltre ad altre che che anche ve ne sono, quali le garanzie funzionali, ma che non toccano questo punto. Il problema era se il Presidente del Consiglio potesse o meno delegare queste funzioni. Certamente pensare che potesse delegarle ad un Ministro

anche con funzioni promiscue, come poi puntualmente è avvenuto. Certamente avere un Ministro o un Sottosegretario con funzione unica è un lusso che un lusso che forse un Governo di cento componenti si sarebbe potuto permettere, ma certamente un Governo di sessanta componenti un lusso del genere non se lo può permettere.

16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*** *(Relazione orale)*